Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Maurizio LUPI dalla carica di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di reggere ad interim il predetto Dicastero. *F.to* Matteo Renzi».

dichiarata aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

La stessa Corte costituzionale, con più sentenze, ha ugualmente dichiarato errato l'utilizzo di questo strumento. mancanza di una maggioranza coesa e quindi dall'obbligo di utilizzare questi strumenti, ovviamente abbinati allo strumento della fiducia, che ormai viene subìto da questo Parlamento, esautorato delle proprie funzioni.

a quello di altri Paesi della zona euro, oltre ovviamente ad una presunta instabilità delle banche popolari. Tutto questo va assolutamente rigettato. È evidente che le banche popolari rispondono chiaramente agli *standard* che la Comunità europea impone. Gli *stress test* operati a livello europeo per le banche popolari sono stati ottimali, dando risposte chiaramente migliori di altre banche, che hanno una struttura di società per azioni. Potremmo sicuramente scoperchiare il vaso di Pandora,

è ormai inesorabile la deriva che vede nel decreto-legge il principale strumento legislativo, soprattutto quando si affrontano questioni complesse e delicate. Anche oggi si discute in quest'Aula di una vera e propria riforma che investe le banche popolari che il Governo presenta come misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Le critiche a questo provvedimento messe in luce da Forza Italia vertono su due diversi profili. Il primo, di carattere politico-costituzionale, è già stato posto all'attenzione di quest'Aula dalla collega Bernini, la quale ha ben spiegato come questo provvedimento non soddisfi nessuno dei criteri costituzionali che riguardano la decretazione di urgenza. Per queste ragioni avremmo voluto che queste misure fossero inserite in un disegno di legge, l'unico strumento idoneo che legittima le funzioni proprie del Parlamento. Il dettato costituzionale secondo cui il Governo esegue ciò che il Parlamento, in rappresentanza della sovranità popolare, decide viene ripetutamente capovolto. Ma questo Esecutivo, è ormai chiaro a tutti, fa un uso assolutamente eccessivo e smodato della decretazione di urgenza e dell'istituto della fiducia, mortificando di fatto costantemente il ruolo delle Camere. E non ci venga a dire il Governo che l'accoglimento di qualche ordine del giorno sparso valga quanto la funzione emendativa del Parlamento. A proposito dell'ordine del giorno del Gruppo di Forza Italia, accolto dal Governo nelle Commissioni industria e finanze e che ricomprende il senso di ben quattro emendamenti, chiedo al sottosegretario Baretta che il testo rechi così com'è stato depositato: «Il Senato impegna il Governo a valutare la possibilità che la trasformazione in società per azioni delle banche popolari avvenga qualora la banca popolare sia quotata in borsa o sia soggetta a vigilanza europea». Quanto al secondo profilo, quello del merito, il nostro giudizio sul provvedimento non è positivo. L'obbligo delle banche popolari di trasformarsi in società per azioni contrasta con una delle caratteristiche principali degli istituti popolari, ovvero lo stretto legame che questi hanno con il territorio. Eliminare questa peculiarità significa cancellare con un colpo di mano una parte importantissima della tradizione e del tessuto bancario italiano come forma Il valore delle banche maggiormente ancorate al territorio sta soprattutto nella loro capacità e sensibilità non solo nel raccogliere numeri, ma anche informazioni qualitative sull'impresa e sull'imprenditore, sul suo *excursus* professionale e personale. Un Paese con milioni di piccole imprese e con grandi differenze tra territori, ha sempre più bisogno di una pluralità di soggetti creditizi solidi che abbiano interesse a capire e soddisfare le diverse esigenze. Il voto capitario, una testa un voto, serviva a preservare la natura di questi istituti bancari in quanto prefigura una finanza costruita non già su logiche di puro profitto bancario, ma intorno ad un'idea forte di coesione territoriale. La *ratio* enunciata dal Governo è quella di creare una nuova *governance* al fine di favorire le aggregazioni interne e di rendere più facile la raccolta di capitali, soprattutto di fronte al rischio di deterioramento dei bilanci. Ma questa impostazione trascura il fatto che i maggiori rischi di crisi finanziaria negli ultimi decenni nascono da banche società per azioni e non da banche a voto capitario. Inoltre, autorevoli economisti osservano che le banche SpA non abbiano tutta questa capacità di reperire in fretta capitali freschi La ricapitalizzazione del Monte dei Paschi da parte del Tesoro con 5 miliardi dimostra che questo istituto bancario, nonostante appunto sia una non è riuscita autonomamente a raccogliere i capitali necessari a superare la crisi che l'ha colpita. Inoltre, ridurre tutti gli istituti bancari all'*unicum* della società per azioni è solo un'iniziativa italiana. Nel panorama europeo esistono diverse forme di banche a voto capitario sopra e sotto la soglia degli 8 miliardi di attivo in Francia, Olanda, Finlandia, Germania e Austria, oltre che in molti Paesi extraeuropei. Vorrei soffermarmi sulla soglia degli 8 miliardi, scelta dal Governo, al di sopra della quale c'è l'obbligo di trasformazione in società per azioni: qual è il criterio che sta dietro questa scelta? Anche la stessa BCE ha selezionato una soglia molto più elevata per l'attivazione della vigilanza bancaria. Non a caso Forza Italia ha proposto che questa stessa soglia, pari a 30 miliardi, fosse applicata come criterio discriminante dell'obbligo di trasformazione. Il provvedimento, come dicevamo disomogeneo, nella seconda parte interviene con misure insufficienti a dare slancio agli investimenti. Viene introdotta una nuova categoria di impresa, la piccola e media impresa «innovativa», a cui vengono riconosciuti i benefici finora riservati alle *start-up*. Le agevolazioni però riguardano soltanto le attività di ricerca e sviluppo, escludendo di fatto tutte le spese relative agli investimenti innovativi orientati al mercato. Inoltre, si prevede un'eccessiva onerosità degli adempimenti burocratici, come le modalità di iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Per nulla convincenti, inoltre, sono tutte le altre disposizioni, che finiscono per agevolare le imprese di maggiori dimensioni, in palese contraddizione con le caratteristiche del del nostro tessuto imprenditoriale. Ancora una volta abbiamo perso l'occasione per attuare una riforma del credito che, finalmente, avrebbe potuto e dovuto dare respiro alle imprese e ai piccoli artigiani che oggi si vedono precluso ogni canale creditizio. abbiamo perso anche l'ennesima occasione per dare slancio agli investimenti.

a quelle la cui dimensione, misurata dal totale dell'attivo di bilancio, non eccede gli 8 miliardi di euro. Rispetto a molte cose che ho sentito, soprattutto nella discussione sulla questione pregiudiziale, va ricordato a quest'Aula

il Fondo monetario internazionale, l'Antitrust e la stessa Commissione europea. Quindi, da questo punto di vista, esisteva un'esigenza oggettiva, anche in relazione al nuovo modello di vigilanza bancaria a livello europeo. Va anche detto, per chiarezza di ragionamento, che non scompaiono le banche di credito cooperativo, che sono 379 nel nostro Paese e sono escluse da questo provvedimento, Governo, giustamente, da questo punto di vista, scelto la strada di sollecitare un'autoriforma delle BCC. Non scompaiono però neanche, come modello,

quelle che superano gli 8 miliardi di attivo contabile. Qui emerge l'altra questione su cui vorrei sollecitare la vostra attenzione. Quando si parla di banche popolari evocando, giustamente, per alcuni versi, la storia, la tradizione, il loro radicamento e il loro ruolo, il loro ruolo, se ne parla come se fossero soggetti dalle dimensioni simili, mentre noi ci troviamo di fronte ad un quadro e a una situazione che negli anni è andata mutando, con una fortissima accelerazione tra

in Italia? Il riferimento, per esempio, è a UniCredit e a Banca Intesa: sono due grandi banche nazionali, presenti in 70 province.

per il sistema delle banche popolari e quindi, in questa prospettiva, si giustifica l'obbligo di trasformazione in società per azioni. Si pone anche un tema di *governance,* su cui però vorrei essere estremamente chiaro. Non sono convinto che esista una forma societaria che metta di per sé al riparo dai rischi legati a una cattiva *governance*. Abbiamo avuto anche di recente l'esempio di società per azioni che hanno avuto problemi e su cui sono in corso indagini della magistratura, alcune alcune delle quali stanno arrivando al giudizio finale. Certamente però il problema riguarda anche le banche popolari - soprattutto le grandi banche popolari - che nel recente passato hanno vissuto episodi gravi.

«causando a volte ingerenze nelle scelte gestionali da parte di minoranze organizzate, in direzioni diverse da quelle dell'utilità per la generalità dei soggetti interessati: soci, risparmiatori, imprese finanziate.

in non pochi casi di gravi difficoltà di banche di ogni forma giuridica, popolari e non. Spesso le difficoltà sono state acuite, anche in misura drammatica, dall'egemonia prolungata e incontrollata di una singola figura o di un gruppo di potere espressione di una minoranza. Nelle grandi popolari il rischio di una deriva di questo tipo è accentuato proprio dalla forma societaria. Nel 2014 alle assemblee delle banche popolari maggiori ha partecipato in media, contando anche le deleghe, poco più di un socio su dieci. Si tratta comunque di svariate migliaia di persone: mobilitarle implica per gli amministratori la necessità di impegnarsi in una vera e propria campagna elettorale, con ovvi rischi di clientelismo».

non prima di aver sottolineato che, per molti aspetti, la soluzione del disegno di legge sarebbe stata preferibile a quella del decreto-legge, perché oggettivamente si interviene su una materia delicata e complessa, come ho provato a ricordare.

Si sarebbe potuto, inoltre, rendere - mi si passi l'espressione «meno appetibili» le popolari, salvaguardando anche alcune peculiarità, perché il rischio di *takeover* ci deve assolutamente preoccupare. Bene, quindi, da questo punto di vista

possano rendere stabile in prospettiva questa limitazione sul modello già utilizzato per la principale banca italiana, che è Unicredit. Inoltre, si sarebbe potuto provare a trovare alcune soluzioni per conservare anche taluni elementi di peculiarità del sistema delle popolari e il loro carattere di radicamento sul territorio. Per esempio, la possibilità di introdurre in statuto, non modificabile se non con maggioranze qualificate successivamente alla trasformazione in Spa, una cinque per cento degli utili per reinvestirli sul territorio; si sarebbe potuto individuare il 20 per cento degli organi sociali votati con voto capitario. In definitiva, l'invito rivolgo al Governo è di accompagnare il percorso di questi 24 mesi, da un lato favorendo certamente i processi di aggregazione e razionalizzazione sotto la guida di Banca d'Italia e dall'altro riconoscendo un valore alla cultura pluricentenaria dalle banche popolari nella prospettiva della nuova vigilanza bancaria europea. con questo provvedimento il Governo intendeva emanare anche un insieme di disposizioni - ordinamentali, finanziarie e fiscali - che incentivassero l'afflusso di investimenti, anche esteri, nel sistema imprenditoriale italiano. Noi abbiamo provato a sostenere le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative tentando di migliorare, con alcune misure, la normativa affinché potesse sprigionare tutte le sue potenzialità producendo ancor più risultati consolidati. Vorrei ricordare all'Assemblea che alla Camera, grazie al Gruppo dei cittadini del Movimento 5 Stelle, si è aggiunto il comma 10*-bis*, che introduce alcuni requisiti di forma per l'atto costitutivo delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati. Nello specifico, si è fatto in modo che l'atto costitutivo e le successive modificazioni siano redatti: per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con firma digitale; secondo il modello *standard* tipizzato dal MISE e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese. Al 1° ottobre 2014 in Italia si contavano 2.655 *start-up* innovative e 31 incubatori certificati; il tasso di crescita di questo ecosistema è tra i pochi a risultare positivo e oscilla tra le 30 e le 40 unità per settimana per quanto concerne le *start-up* innovative. dicembre 2014 il numero di *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese è di 3.179 unità, in aumento di ben 549 unità rispetto a fine settembre. Le *start-up* sono lo 0,21 per cento del quasi 1,5 milioni di società di capitale italiane. Il capitale sociale delle *start-up* è complessivamente di 153 milioni di euro, che corrisponde in media a circa 48.000 euro a impresa. Il capitale medio è in aumento di quasi il 20 per cento rispetto al terzo trimestre. Dal punto di vista settoriale, quasi il 73 per cento delle *start-up* innovative fornisce servizi alle imprese, il 18 per cento opera nei settori dell'industria in senso stretto e il 3,8 per cento nel commercio. I principali attori sulla scena italiana dell'innovazione segnalano la difficoltà nel fare impresa, in particolar modo in settori che richiedono un'elevata specializzazione tecnica. Un grave problema è la scarsa intenzione degli investitori privati di elargire finanziamenti, questo a causa della scarsa credibilità del sistema Paese che trova le sue radici profonde nell'eccessivo costo del lavoro e nell'elevata tassazione, nell'incertezza del diritto e della giustizia e nell'insormontabile burocrazia. Le *start-up* con una compagine societaria a prevalenza femminile sono il 12,5 per cento del totale. Quelle a prevalenza giovanile (*under* 35) sono il 26 per cento del totale: una quota superiore a quasi quattro volte quella delle società di capitale giovanili. In valore assoluto, Milano è la provincia che ospita il numero maggiore di *start-up* innovative, 466; seguono Roma, Torino, Trento e Napoli. Se però si considerano tali valori in rapporto al numero di società di capitali presenti nella Provincia, Trento è prima in classifica con 103 *start-up* ogni 10.000 società di capitali, mentre Milano è molto distante con un indice pari a 29. Complessivamente le *start-up* innovative hanno registrato una produzione pari a quasi 213 milioni di euro nel 2013. Una delle caratteristiche peculiari delle *start-up* innovative è l'elevato grado di immobilizzazione dall'attivo patrimoniale: il rapporto è pari al 30,5 per cento ed è cinque volte il rapporto medio delle società

La struttura finanziaria delle *start-up* innovative è relativamente migliore di quella delle società di capitale. Situazione inversa per le *start-up* in utile, che hanno una situazione finanziaria peggiore della media delle società di capitale. A conti fatti, per ogni euro di produzione le *start-up* innovative generano in media 13 centesimi di valore aggiunto, un dato più basso di quello delle società di capitali (20 centesimi). Limitatamente alle imprese in utile, le *start-up* generano invece più valore aggiunto delle società di capitali (32 centesimi contro 22). Per tutti questi motivi volevamo migliorare, ripeto, con alcune misure la normativa a sostegno dell'ecosistema della *start-up*, a partire dalle modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali *online*. Abbiamo proposto: l'abolizione del contributo minimale INPS per i soci amministratori di *start-up* innovative; il contributo ammonta a circa 3.600 euro l'anno. Lo Stato ipotizza un reddito minimo e, quindi, fissa una soglia minima di contributi. Ma le *start-up* possono avere anche reddito zero per quattro o cinque anni, perché l'obiettivo delle *start-up* non è quello di generare reddito in fase iniziale. Abbiamo proposto l'esenzione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità, che è un onere burocratico che racchiude in sé informazioni di carattere fiscale. Abbiamo proposto la gratuità della prima vidimazione dei libri sociali. Si trattava di poche centinaia di euro, ma sarebbe stato un aiuto. Abbiamo proposto l'esenzione dal pagamento di concessione governativa per il primo anno primo anno e la realizzazione di spazi di *coworking* da destinare alle PMI innovative attraverso la riqualificazione di patrimonio immobiliare pubblico al fine di promuovere la nascita di nuove *start-up* Lo Stato poteva promuovere l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, per istituire spazi di *coworking*. Con queste proposte emendative intendevamo lanciare un grande segnale al Paese, ai nostri giovani all'estero e agli investitori, che investono da noi, che in Italia è più facile e conveniente fare innovazione. Ma evidentemente abbiamo profonde e differenti visioni su come migliorare le potenzialità del nostro Paese. Anzi, a dire il vero, a voi le potenzialità del Paese interessano, ma solo ed esclusivamente per spolparlo fino al midollo.

i segnali positivi che arrivano dalla nostra economia sono incoraggianti anche se la strada è ancora lunga. I recenti dati dell'OCSE ci dicono che il nostro Paese può agganciare la ripresa economica: l'Italia è passata da uno stallo sulle riforme a un passo ottimale di riforme, e per questo siamo più positivi sulle prospettive future, ci dicono dall'organizzazione. Per il Paese, aggiungono, ci sono opportunità anche grazie a un contesto migliore. Per questo occorre spingere sull'acceleratore in direzione delle riforme che Governo e Parlamento esaminano in questi mesi. Bisogna fare tutto quanto è necessario per rafforzare questi impulsi positivi e solidificare la ripresa, quindi insistere sul programma di riforme strutturali. In questo contesto e con queste premesse intervenire sul sistema bancario è un elemento fondamentale. Per questo è importante il provvedimento di cui discutiamo. Le misure introdotte in questo decreto-legge sono determinanti perché volte al rafforzamento del sistema bancario, adeguandolo allo scenario europeo ed internazionale. Il provvedimento sulle banche popolari e gli investimenti riforma un comparto fondamentale della nostra economia, in modo da renderlo più solido al fine di rafforzare l'impegno a sostegno degli investimenti e dell'*export* per le nostre imprese. Un intervento, quello sulle banche popolari, non punitivo, il cui obiettivo è quello di lavorare per modernizzare questi istituti, che hanno tutte le caratteristiche delle banche tradizionali, ma che conservano una forma di *governance* che in alcuni casi non ha dato buona prova di sé. La trasformazione delle banche popolari in società per azioni risulta, dunque, centrale di fronte ai cambiamenti bancari nello scenario *post*-crisi. Il decreto-legge tiene conto del ruolo che questi istituti hanno sul territorio, un ruolo che le ha viste molto spesso garantire giustizia sociale, soprattutto - non dimentichiamolo Lo stesso presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, ha recentemente spiegato che questo decreto-legge va nella giusta direzione. Rimuovere ostacoli ed incrostazioni normative è il senso dell'intervento sulle banche popolari. Mi preme però soffermarmi sul capitolo che questo provvedimento dedica alle piccole e medie imprese. Si tratta di una parte importante e non secondaria, ingiustamente oscurata dalle polemiche sulle banche popolari,

un provvedimento che dà un impulso forte anche allo sviluppo di piccole e medie imprese innovative, con una serie di norme che creano condizioni favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle PMI innovative permettendo di dare un contributo rilevante alla crescita economica e all'occupazione, in particolare a quella giovanile e specializzata. È un provvedimento che rende il nostro sistema sempre più attrattivo, attrattivo per le imprese innovative, capaci a loro volta di attrarre investimenti finanziari per tale settore e di essere competitivo sui mercati internazionali. Importante è inoltre il capitolo che punta a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana con Cassa depositi e prestiti, che erogherà il credito anche tramite SACE. Viene quindi autorizzato l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione separata di Cassa depositi e prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese.

le imprese che svolgono attività d'impresa da non più di cinque anni, mentre attualmente il limite è di 48 mesi. Per la gestione degli atti inerenti alle piccole e medie imprese innovative viene fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Si prevede, inoltre, che potranno usufruire degli incentivi all'investimento

un portale nel quale saranno indicati tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati, diretti ed indiretti, a favore delle piccole e medie imprese innovative È potenziata, inoltre, l'operatività del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese: il limite stabilito del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione sarà solo per la garanzia diretta. Si rafforzeranno poi le procedure di recupero dei finanziamenti per i quali è stata escussa la garanzia del fondo e diverrà più semplice trasferire il proprio conto corrente e aprire un conto transfrontaliero. L'operatività del Fondo verrà estesa alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento, diverse dal rilascio di garanzia, verso soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. Con una delibera del CIPE, inoltre, dovranno essere emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione. Molto importante, colleghi, è il fatto che verrà riconosciuta priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il consiglio di gestione del Fondo dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalle richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta. inoltre particolare apprezzamento l'articolo 7 del decreto-legge, che dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, avente sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. L'obiettivo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese che siano comunque caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate alcune modifiche concernenti l'ambito di operatività, le finalità, i sottoscrittori e le modalità operative della società. In particolare, si è ampliato l'ambito operativo della società, eliminando l'esclusivo riferimento alle imprese industriali tra quelle per il rilancio delle quali la stessa società potrà intraprendere iniziative; si specifica che la società dovrà favorire processi di consolidamento sia industriale che occupazionale. Infine, ma non per importanza, segnalo la norma che obbliga gli istituti di credito a trasferire, senza costi, i conti correnti dei clienti entro dodici giorni lavorativi; un segno di attenzione per famiglie e consumatori. Signor Presidente, chiudo l'intervento dicendo che questo provvedimento risulta essere un altro tassello importante per questo Governo e per le forze responsabili del Parlamento che si aggiunge ad un processo di riforme - come menzionato all'inizio - già in atto. Un processo di rinnovamento e di riforme

Signor Presidente, è evidente a tutti che la parte più rilevante di questo decreto-legge è quella relativa alla trasformazione delle banche popolari

Nel metodo, perché viene attuata con il solito sistema "renziano" dei decreti-legge e della fiducia posta all'ultimo momento,

Al Senato della Repubblica, quindi, viene concesso un solo giorno per la discussione di questo provvedimento e di fatto si impedisce la manovra emendativa,

di urgente, ma contengono temi molto eterogenei al loro interno. A Renzi, però, tutto è concesso, mentre in altre situazioni, nei confronti di altri Governi, si sarebbero sollevati gli strali del Presidente della Repubblica quelli che ci hanno governati in questi ultimi decenni, e vi sarebbe stata la levata di scudi di molti autorevoli costituzionalisti e intellettuali, dei giornali e di quant'altro. Nella realtà dei fatti, però, a Renzi tutto è permesso, come pure questa riforma

dall'Unione europea, come spesso ama dire il Presidente del Consiglio. Non ce lo chiede l'Europa, in sostanza, perché questo tipo di istituti bancari, a carattere mutualistico e cooperativo, esiste in tutta Europa, come ad esempio in quella Germania spesso utilizzata come modello di sviluppo economico. noi facciamo una scelta opposta ed in controtendenza, decidendo la cancellazione delle banche popolari, la loro trasformazione, coattiva ed obbligatoria, in società per azioni e lo snaturamento della loro funzione, anche sociale, per l'economia dei nostri territori. Tengo a ricordare che le banche popolari rappresentano una ricchezza una ricchezza per l'accesso al credito del sistema delle piccole e medie imprese soprattutto del Nord Italia e del mio Veneto, poiché hanno permesso l'accesso al credito alle famiglie ed alle piccole industrie, soprattutto in questi ultimi anni di crisi, con una proporzione di disponibilità nei confronti di questo tessuto economico ben superiore alle grandi banche, che hanno come fine sociale non solo un effetto mutualistico e cooperativo nei confronti dei propri soci e del territorio, ma finalità soprattutto finanziarie e di capitalizzazione del reddito. Secondo la nostra visione delle cose,

della democrazia e delle regole del libero mercato che evidentemente hanno il Partito Democratico e il suo presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ed è evidente a tutti che il suo modello di democrazia non è certamente il nostro: fa riforme in cui si dice che vengono cancellate le Province, ma di fatto l'unica cosa che viene cancellata è la rappresentanza democratica

il famoso Porcellum, tanto vituperato dal Partito Democratico - ma si fa sostanzialmente un Porcellum 2, in cui tre quarti dei nuovi eletti saranno nominati dai capipartito e, in particolare per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, dal capopartito che lui continua ad essere, pur essendo Presidente del Consiglio. Si tratta quindi di una visione democratica che a noi non piace e che non condividiamo: di fatto, viene esautorato il potere popolare di scelta dei propri rappresentanti e anche in questa scelta vediamo lo stesso atteggiamento e lo stesso rischio.

ed è quindi inaccettabile questo tipo di trasformazioni nell'interesse di pochi. Questa riforma sta passando nel silenzio, come tutte le cose negative che sta facendo l'attuale Governo purtroppo ha creato un sistema in cui è tutelato dai grandi gruppi di potere e dalla grande informazione, in cui sono poche ormai le voci di dissenso nei confronti del Presidente del Consiglio. Ma una voce rimarrà sempre in questo Parlamento e sul nostro territorio, la voce libera della Lega Nord e dei suoi rappresentanti, che, al di là delle finte riforme del Governo Renzi, cercherà di spiegare ai cittadini quello che sta avvenendo in questi palazzi a totale dispregio della democrazia e degli interessi del Paese.

affrontiamo oggi in quest'Aula la riforma del sistema delle banche popolari, un provvedimento di cui sia Banca d'Italia, che il Fondo monetario e la Commissione europea auspicavano l'avvio. Il testo all'esame prevede che le banche popolari detentrici di un attivo consolidato superiore a 8 miliardi di euro - e ne sono state identificate dieci - debbano attivare, entro i 18 mesi dal regolamento attuativo di Banca d'Italia, una tra le seguenti azioni: la riduzione dell'attivo, riportandolo sotto la soglia degli 8 miliardi; la trasformazione in società per azioni ordinarie, abbandonando così la *governance* storica basata sul voto capitario, oppure ancora la scelta di arrivare alla liquidazione; in caso di inadempienza la legge dell'assemblea dei soci la Banca d'Italia potrà agire per ottenere la revoca della licenza bancaria. È una lunga storia quella delle banche popolari, che trova le sue radici nella tradizione cooperativistica socialista e dell'associazionismo cattolico. Uno strumento mutualistico dal quale contadini, artigiani e piccoli imprenditori uniti dalla convivenza su un territorio trovarono una risposta al bisogno di credito e di una gestione della sua erogazione vicina alle loro realtà economiche e sociali, ai loro bisogni. Un problema, quello dell'erogazione e del bisogno di credito, che ancora oggi permane e sul quale ancora molto lavoro dobbiamo spendere. Il sistema delle banche popolari si è poi modificato nel tempo e mi scuso per l'abbreviazione di una storia così importante, della quale sarebbe utile conservare negli atti e statuti che accompagneranno la prossima trasformazione ed anche in quella fetta di sistema che permarrà, i valori della cooperazione, del mutualismo e del collegamento, inteso nella sua accezione positiva, con le comunità locali. Le modifiche che il tempo ha generato nel sistema delle banche popolari quali l'ingrandimento del giro d'affari dovuto sia alla naturale crescita, che alle necessità di vigilanza e di sicurezza del credito, lo sconfinamento dalle realtà territoriali che le avevano generate ed anche l'uniformità dell'offerta dei prodotti, appiattita alle proposte di un mercato dove la ricerca e l'esclusività di un servizio hanno brevissima durata, generano oggi una anomalia nel settore del credito cui la riforma mette mano. Anche la *governance* storicamente caratterizzata dal voto capitario, una testa un voto, ha messo in luce tutte le tante criticità che oggi vanno risolte, ad esempio la trasparenza nella raccolta delle deleghe in assemblea e nel trasferimento delle azioni per le banche non quotate, la scelta del *management* oltre all'abitudine - rilevata in alcune realtà - del formarsi di dinastie di amministratori e al superamento dell'autoreferenzialità. Partiamo quindi da queste osservazioni e da questi limiti, sapendo che il modello del voto capitario era stato pensato a tutela del patrimonio delle banche popolari quale frutto di una specifica collettività: esso impediva infatti acquisizioni speculative o scalate da parte di altre banche o privati. Questa riforma cambierà quindi profondamente la loro struttura ed impostazione. Le banche popolari, alcune delle quali sono in crisi e sono alla ricerca di nuovi capitali, potranno rientrare in processi di fusione o aggregazione esattamente come successo per altri istituti di credito in questo settore. ritengo positivo accompagnare questo momento di riorganizzazione limitando l'esercizio del diritto di voto al 5 per cento del capitale sociale nei primi due anni dalla trasformazione in società per azioni, per evitare appunto questi effetti speculativi. Fatta questa premessa, voglio oggi riportare la lettura che in Commissione lavoro abbiamo dedicato a questo provvedimento, che non si occupa solo di riforma delle banche popolari, ma anche di misure per la piccola e media impresa innovativa, apprezzando le opportunità di consolidamento del lavoro dipendente altamente qualificato. Questo provvedimento fa infatti nascere la nuova categoria delle PMI innovative, che potranno accedere alla maggior parte delle semplificazioni e agevolazioni oggi previste per le *start-up*, tipologia di impresa nata da non più di quattro Il provvedimento fissa i requisiti per rientrare nella categoria delle piccole e medie imprese innovative ed essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese. Oltre ad alcune caratteristiche di bilancio e societarie, è richiesto che ricorrano almeno due dei tre requisiti indicati e, tra questi, la presenza di personale (dipendenti e consulenti) altamente qualificato, presenza che viene stabilita in percentuali puntuali rispetto alla forza lavoro e variabili a seconda che si tratti di dottori o dottorandi di ricerca o di laureati con esperienza triennale certificata di ricerca oppure con laurea magistrale. Ritengo sia un'opportunità importante di stabilizzazione del lavoro altamente qualificato. Conseguenze diverse invece sul versante lavoro per la parte relativa alla riforma delle banche popolari. Abbiamo infatti rimarcato in Commissione come il processo riorganizzativo che coinvolgerà il sistema delle banche popolari dieci banche attualmente identificate sulla base dei numeri e tutto il sistema che da questo processo potrebbe essere coinvolto) metterà a rischio il livello occupazionale dei dipendenti bancari del comparto. Sono 60.000 gli addetti impiegati oggi e le previsioni di Assopopolari stimano nel 20 per cento i posti a rischio. La categoria del credito ha fino ad oggi superato molte ristrutturazioni grazie a buone coperture garantite da accordi bilaterali, mancando gli ammortizzatori pubblici utilizzati per le altre categorie di lavoratori. Saranno quindi necessari sia un puntuale monitoraggio dei processi riorganizzativi che azioni di accompagnamento nella direzione di unificare le misure pubbliche e di arrivare a strumenti bilaterali sulla base di accordi tra le parti.

Lo si è visto in modo chiarissimo nelle privatizzazioni delle grandi aziende statali e nelle varie riforme, reali o annunciate, della pubblica amministrazione. Nessuno può negare che il sistema delle partecipazioni statali andasse ampiamente rivisto e corretto: la sua quasi completa dismissione ha però avuto l'unico effetto di creare nuovi monopoli e nuove e più gravi fonti di inquinamento della vita pubblica. Nessuno può negare che l'intero comparto pubblico vada migliorato e reso più efficiente. I continui tagli, spesso giustificati da una campagna di demonizzazione dei pubblici dipendenti tutti indistintamente dipinti come incapaci e fannulloni - hanno però avuto l'unico effetto di peggiorare la qualità dei servizi essenziali o di renderli addirittura inaccessibili alle persone comuni. comuni. Sospetto che qualcosa del genere stia ora avvenendo anche con la riforma delle banche popolari. Vi sono stati certamente degli abusi nella gestione di alcune di esse. Questi fenomeni, però, possono e devono essere corretti con gli strumenti che già che già esistono: con l'applicazione, cioè, dei principi del diritto bancario, del diritto civile e del diritto penale. Purtroppo, invece, ancora una volta si getta il bambino con l'acqua sporca. O meglio, l'acqua sporca è presa a pretesto per gettare il bambino. A dispetto di tutti gli abusi, deve infatti essere chiaro che le banche popolari hanno svolto un ruolo molto positivo nell'economia nazionale. Il loro legame con il territorio ha permesso per anni l'accesso al credito di aziende piccole o artigiane, che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a finanziarsi. Con la loro stessa esistenza, esse hanno alimentato, come ricorda in un recente articolo «Avvenire», quella biodiversità economica che, accanto a quella culturale, è stata il vero tesoro di un Paese ricco delle sue diversità. Questo ora non avverrà più. Una cosa, infatti, deve essere chiara. Il provvedimento che obbliga le banche popolari a trasformarsi in società per azioni, rinunciando così alla loro natura cooperativa fondata sul voto capitario (una testa vale un voto), segna la fine di questa originaria espressione della nostra economia. Da ora in poi comanderà chi ha più azioni. Si cercherà il profitto dove si riterrà opportuno e nelle forme che più si riterranno opportune. In tal modo il carattere locale e territoriale delle banche popolari verrà meno. Nulla impedirà alle banche popolari, così snaturate, di dedicarsi alla speculazione, giocando sui derivati e sugli altri marchingegni della finanza creativa. Nulla impedirà che capitali accumulati col lavoro e le fatiche delle comunità locali finiscano in mano a persone pronte a gestirli sulla base interessi del tutto estranei a quelli di queste località. È questo quello che vogliamo? La vicenda del Monte dei Paschi di Siena che, dopo secoli di gloriosa esistenza come banca locale, si è trovata sull'orlo del fallimento nel momento in cui ha deciso si internazionalizzarsi, dovrebbe averci insegnato qualcosa. Purtroppo, in un mondo in cui, come ha dimostrato Thomas Piketty sulla base di dati difficilmente contestabili, la principale fonte di arricchimento e potere si sta rapidamente spostando dalla produzione alla rendita: la stessa presenza di soggetti finanziari legati all'economia locale viene presentata come un'assurdità arcaica. È stato affermato che con questa riforma si toglieranno le banche ai signorotti locali; dubito che questo sia vero: la storia italiana dimostra che i signorotti locali riescono quasi sempre a farla franca, magari cambiandosi d'abito e mettendosi al servizio di nuovi interessi. Ritengo invece più probabile che ai vecchi signori se ne aggiungano di nuovi, nazionali ed internazionali, internazionali, ancora peggiori, in quanto indifferenti alle sorti ed ai destini del nostro Paese. A farne le spese sarà, ancora una volta, Pantalone.

Che cosa sono le banche popolari oggi in Italia? Sono banche esattamente come le altre, solo che hanno diverse peculiari regole di funzionamento, quali per esempio il gradimento dei soci attuali rispetto ai nuovi. La regola del gradimento comporta che, se una persona vuole comprare azioni di una banca popolare ed esercitare i diritti che da quell'acquisto derivano (voto in assemblea, ispezione dei libri sociali, impugnazione delle delibere assembleari), deve chiedere il permesso a quelli che sono già Poi, a prescindere dal numero di azioni detenute, ogni socio ha un solo voto. Ancora, nessun socio può avere più dell'uno per cento del capitale, fatta eccezione per i fondi d'investimento, che non hanno limiti di azionariato, ma che comunque non possono esprimere più di un voto. Una volta, le banche popolari avevano il carattere della mutualità, che derivava loro dalla forma cooperativa della società. Se questo spirito filantropico e mutualistico sussista ancora nelle società cooperative in generale, è tutto da dimostrare, vista la logica operativa della stessa Legacoop e di molte sue associate. Certo è, però, che le banche popolari, oggi, hanno ampiamente perso ogni caratteristica di mutualità. Nel Testo unico del 1993 un vincolo di destinazione a fini sociali o di beneficenza di una quota degli utili per le banche popolari manca del tutto. In sostanza, le banche popolari sono banche in cui l'elemento personale conta molto di più di quello patrimoniale e questo - se mi è concesso - è una contraddizione in termini. La banca popolare non è un ente di beneficenza o un'organizzazione *no profit*: è un'impresa che cerca utili. È un'impresa, però, in cui gruppi d'amicizia, cordate di persone, sindacati di dipendenti contano molto di più delle energie economiche e finanziarie che vi profondono. Il Governo sostiene che questo sistema, sopra gli otto miliardi di attivo - badate: otto miliardi - deve finire. Personalmente, sono d'accordo. Le banche cooperative di credito, che sono volte a fare credito ai soci, restano intatte, così come le banche popolari, la cui massa attiva (cioè i crediti concessi) si collochi sotto gli otto miliardi, restano al loro posto. Quelle che invece si dovranno trasformare in banche ordinarie, con la forma di società per azioni, hanno un attivo superiore agli otto miliardi. Che la gestione personale capitaria delle banche popolari sia un presidio alle scorribande di personaggi disinvolti è poi smentito dalla storia recente della Banca popolare di Milano, che solo tre anni fa è stata investita da uno scandalo di vaste proporzioni (le indagini mi risultano concluse nel marzo 2014). Di fatto, l'ex presidente di quella popolare è stato accusato di avervi stabilito una "struttura parallela" di concessione del credito che favoriva i politici di Milano, come - tra gli altri - esponenti che sono ancor oggi in Parlamento. Egli fu accusato di avere un rapporto privilegiato con uno strettissimo collaboratore dell'allora ministro Tremonti e con molti politici, per cui il credito non veniva fatto a chi meritava, ma a chi era amico della cricca. La Popolare di Milano risulta anche aver dato ingenti finanziamenti alle società che gestiscono le *slot machine*, che non è propriamente il piccolo e ingegnoso artigianato locale. non dico che nelle banche ordinarie non succedano queste cose, ma dico che la struttura delle banche popolari non è stata garanzia che non succedessero. Vengo all'obiezione più rilevante che viene mossa alla riforma contenuta nel decreto-legge n. 3: le grandi banche commerciali avrebbero una struttura e un'organizzazione insensibile alle esigenze della morfologia produttiva italiana, cioè il tessuto a rete di piccole e medie imprese. Si sostiene da varie parti che le piccole e medie imprese trovano poco ascolto nelle procedure standardizzate e rigide delle grandi realtà bancarie, giacché queste rispondono all'ottica del profitto su scala internazionale e secondo il profilo marcatamente finanziario dell'economia globale, e trascurano i bisogni dell'economia reale radicata sul territorio. Esponenti delle banche popolari sottolineano che, nel periodo 2008-2013, le banche commerciali avrebbero contratto il credito del 16 per cento, mentre le popolari lo avrebbero aumentato del 4,9. Questi dati percentuali, in realtà, non sarebbero decisivi, giacché bisogna sempre considerare i dati di partenza, che non vengono esposti. Se, per esempio, le grandi banche partivano da enormi esposizioni verso le imprese all'inizio del periodo di crisi, aver contratto nel complesso gli impieghi del 16 per cento non significa, di per sé, che abbiano chiuso i rubinetti del credito. Osservo tuttavia che, tra le banche popolari che verranno interessate dal provvedimento, ci sono due istituti di credito che hanno rispettivamente una massa attiva di 126 miliardi (il Banco (il Banco Popolare, cioè la banca derivante dall'aggregazione di molte banche popolari quali, tra le altre, la Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero e la Popolare di Lodi, poi Banca Popolare Italiana, quella di Fiorani, non proprio un bell'esempio) e di 124 miliardi (la UBI Banca). Non mi sembrano, quindi, realtà bancarie particolarmente legate a specificità territoriali. L'impressione è, invece, che la progressiva concentrazione delle banche popolari abbia seguito una traiettoria assai simile alle banche commerciali, le cui caratteristiche, invece, i critici del decreto-legge censurano. Inoltre, occorre ribadire che non tutte le banche popolari vengono costrette alla trasformazione, ma solo quelle di grandi dimensioni. Se vi è una sperimentata attitudine delle piccole banche popolari a finanziare le iniziative imprenditoriali del territorio, ebbene questa attitudine è conservata dal limite degli 8 miliardi e dalla permanenza delle banche di credito cooperativo. Le banche popolari che vengono indotte a trasformarsi in società per azioni sono quelle che hanno, ciascuna, sportelli nel sportelli nel 60 per cento del territorio del Paese ed è, quindi, un po' difficile che si atteggino a "banchetta dell'angolo della strada", come il fornaio. Da ultimo, ma non per importanza, sottolineo il tema della vigilanza bancaria europea. L'integrazione in Europa porta anche l'esigenza che parametri uniformi di vigilanza (cioè il controllo del rispetto delle regole da parte di un'autorità indipendente) siano rispettati. Uno di quei parametri è il patrimonio bancario, che deve essere posseduto per far fronte ai rischi dell'attività, giacché - scusate l'ovvietà - fare credito non è esattamente come vendere camice. Noi sappiamo che le banche popolari in Italia hanno crediti deteriorati in misura percentuale maggiore della media delle banche italiane e, quindi, hanno recentemente avuto bisogno di misure di rafforzamento patrimoniale, che è stato complicato attuare con un *management* inamovibile, perché deciso da organi societari in cui vige il principio: una testa, un voto. In conclusione, l'articolo 1 del decreto-legge mi trova sostanzialmente d'accordo. Quanto, poi, all'articolo 2, sulla portabilità del conto corrente, sono pienamente soddisfatta, giacché si tratta di una mia personale battaglia. Per questi motivi, non sono propensa a sottoscrivere le perplessità che sono state espresse e annuncio il mio voto favorevole. Signor Presidente, è da vent'anni che si discute delle banche popolari perché una riforma andava fatta. proprio perché il discorso è delicato e va ad incidere pesantemente sull'economia reale, la riforma non andava fatta con un decreto-legge. L'unica urgenza che sembra palesarsi leggendo questo atto del Governo è l'impossessarsi, nell'immediato, dei risparmi degli italiani, entrando a gamba tesa nel libero associazionismo e portando avanti la guerra dei capitali. Questo decreto-legge viola, a livello giuridico, gli articoli 2, 3, 18, 41, 45 e 47 della Costituzione. Dettagli! praticamente, di un esproprio miliardario. Non ha alcun senso a livello economico. Ricordo, infatti, che 163 economisti hanno firmato un appello per fermare questa riforma e Rete Italia ha detto, in audizione, che questa è un'operazione molto pericolosa, che mette a rischio il finanziamento delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Infatti, le banche SpA sono più propense a fare *trading* finanziario, piuttosto che credito, perché il credito rende troppo poco per un mercato così competitivo. Infatti, le società per azioni hanno una minore intensità di credito sul totale dell'attivo. Si passa, per dieci banche, da voto capitario a quota azionaria e si inserisce una modifica al diritto di recesso anche in deroga alle leggi. Quindi, si va ad incidere su un sistema che era di democrazia economica. Perché, invece, non preoccuparsi dell'altro sistema bancario, che ha provocato la crisi finanziaria globale e che, a differenza delle banche cooperative, è a rischio sistemico? State cambiando l'equilibrio del sistema bancario italiano, ancora una volta, per salvare le banche - le banche SpA - e dare loro la possibilità di appropriarsi dei capitali sani delle popolari. Diciamolo: queste dieci nuove banche SpA salveranno le banche dei vostri amici, che come Stato non siete riusciti a salvare, aprendo inoltre alla speculazione il risparmio italiano, che ha un mercato ancora molto ricco - parliamo di quasi 1.000 miliardi di euro - su cui in molti vogliono mettere le mani. La mafia c'è riuscita, entrando nell'economia reale del Nord, perché ha capito che il vero *business* ormai è il PIL privato e non più quello pubblico. Voi lo fate in parte con questo decreto-legge, ma ho già detto in questa Aula che lo Stato è diventato la peggiore delle mafie. in esame non si parla solo di riforma delle popolari, ma si mette di nuovo mano anche al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ampliando ancora una volta la platea offrendo la garanzia dello Stato anche ad operazioni già deliberate. Che cosa stiamo garantendo? Contratti già sottoscritti, che non conosciamo.

Il provvedimento cerca inoltre di attirare capitali esteri in Italia. Ma trattando questo argomento, sottosegretario Baretta, dimentica sempre che i capitali esteri non saranno mai investiti in Italia se non si risolve il problema della corruzione, che fa lievitare i costi, e senza una certezza fiscale e tributaria. che, negli ultimi 12 mesi, ci sono state quattro modifiche della disciplina tributaria per ogni giorno lavorativo: come pensate che dall'estero possano investire con queste condizioni di incertezza?

iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà. finestra") *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci avviamo a convertire in legge merita che si manifestino in quest'Aula un commento e una speranza. il commento: la trasformazione forzosa in società per azioni delle popolari maggiori non è di per sé un errore - anzi - ma le modalità con cui viene fatta suscitano diffuse riserve, che condivido.

le grandi popolari non sono più cooperative perché slegate ormai dai territori d'origine. Ciò è giusto, ma è ancor più giusto dire che tutte le popolari sono cooperative spurie. A differenza delle cooperative propriamente dette, esse pagano dividendi e possono, se credono, distribuire il patrimonio tra i soci. Lo scambio mutualistico è pressoché inesistente. Ma allora - dico io - perché limitare la trasformazione in società per azioni alle sole popolari di maggior dimensione? E se è la dimensione a minare la natura cooperativistica di queste aziende e non le regole sul patrimonio sul patrimonio e sugli utili, perché limitarsi a trasformare in società per azioni le cooperative di credito e non anche altre grandi cooperative di rilievo nazionale e internazionale nei settori del consumo e della produzione? non mi auguro ciò ma, proprio perché non me lo auguro, spero che, nella replica, il Governo, nel quale siede un alto esponente delle cooperative, come il ministro Poletti - rappresentato qui dal vice ministro Baretta, che viene dal sindacato faccia chiarezza su questi punti. E non vorrei non accadesse perché, non di rado, la logica finisce dove inizia la politica. Vi è Se la dimensione è il criterio scelto dal Governo, come si stabilisce la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di diventare società per azioni? L'Unione bancaria europea fissa in 30 miliardi il limite minimo per essere considerate banche di rilievo sistemico. Un criterio non troppo logico, ma comunque equitativo, avrebbe potuto essere stabilire la soglia europea e comunque la soglia qualitativa dell'essere quotate per trasformarsi in società per azioni. Mi chiedo: perché fare del *gold-plating*, o, per uscire dal gergo, perché fare i "pierini", e dire invece 8 miliardi? Qualcuno ha sospettato, che in tal modo, si potevano infilare nel lotto le due popolari venete non quotate e la Popolare dell'Etruria, quotata ma disastrata, con quella di Bari come foglia di fico finale. Non mi iscrivo Il problema principale è dato dagli effetti che questo decreto-legge avrà sugli assetti di controllo delle grandi popolari una volta trasformate in società per azioni. Il voto capitario rendeva non contendibili le popolari, se non a caro prezzo, come accadde per la Banca agricola mantovana Banca cooperativa di Imola, scalate con successo, l'una dal Monte dei Paschi e l'altra dalla CariRavenna. Non è questa la sede per discutere dei vantaggi della contendibilità elevata a *totem* per il sistema finanziario, che opera nei tempi brevi, e degli svantaggi per il sistema industriale, che lavora sui tempi lunghi. Sarebbe forse il caso che i partiti - e anche il mio trovassero il modo di ragionarne, dati alla mano. Ma stiamo al tema. Senza più voto capitario, le popolari diventano contendibili, avendo esse compagini azionarie assai frazionate. La Banca d'Italia ritiene che, in tal modo, possano fare più facilmente gli aumenti di capitale che la vigilanza europea richiederà. Il direttore generale Rossi ha riconosciuto in audizione alla Camera che le popolari oggi hanno un patrimonio di miglior qualità analogo a quello delle banche SpA, ma ricorda come a questo risultato si sia arrivati *in extremis* e in virtù delle pressioni della Banca d'Italia. Sempre Rossi ha rammentato come i crediti deteriorati delle maggiori popolari siano pari al 18 per cento degli impieghi - due punti in più della media del sistema - e come il grado di copertura dei fondi rischi sia di poco superiore al 30 Personalmente, avrei completato il quadro statistico ricordando che i crediti deteriorati sono espressi al lordo e che, nel paragone con la media delle 13 banche vigilate dall'Europa, le popolari maggiori non vanno poi così male (c'è un punto di differenza); come il *coverage ratio*, a cui abbiano fatto prima riferimento, sia basso soprattutto in una delle popolari maggiori, quella che però ha i mezzi propri più alti, superiori, in proporzione, a quelli di Unicredit e di Intesa San Paolo. E soprattutto, avrei ricordato che la patrimonializzazione delle banche non è un dato assoluto, bensì un rapporto tra il patrimonio netto e gli attivi ponderati per rischio e che, sotto questo profilo, le banche società per azioni più grandi si sono sistemate sia facendo aumenti di capitale sia, soprattutto, tagliando i prestiti alla clientela, mentre le popolari maggiori hanno dato più fiducia e, quindi, hanno imbarcato più perdite reali e potenziali sui crediti. Giusto per dare anch'io tre numeri, e completare il quadro svolto dalla senatrice Ricchiuti, dico che, tra il 2003 e il 2013, le popolari hanno aumentato del 117 per cento i loro prestiti, anno dopo anno; le banche di credito cooperativo (BCC) hanno aumentato i loro crediti alla clientela del 91 per cento, mentre le SpA, che negli ultimi anni li hanno pesantemente tagliati, li hanno aumentati nel decennio soltanto del 38 Fatico, quindi, a seguire - è una mia debolezza, altri sono più bravi di me - la logica secondo cui, in tempi di recessione, il lunedì si invitano le banche a dare più credito alla clientela, e il martedì le si rimprovera perché, dandolo, hanno avuto più sofferenze. L'esperienza di trent'anni mi suggerisce qualche altro dubbio. Essere contendibili vuol dire essere scalabili. Ma una volta scalati, si diventa non più contendibili:

fu proprio Deutsche Bank a dare il via alla speculazione internazionale contro il debito pubblico italiano. Ce lo siamo dimenticati? Io no. Capisco che questa grande banca tedesca, imbottita di derivati (ha il *record* europeo in materia),

è stata scalata e il nuovo padrone l'ha spolpata. Il Crediop è stato preso da Dexia ed è andato anche peggio. La vigilanza si è dimostrata impotente a far sì che il cambio di proprietà facesse bene ai conti. Quali garanzie abbiamo che la storia non si ripeta? Delegare tutto alla vigilanza europea, occhiuta sulle attività bancarie di tipo commerciale (le nostre) e assai indulgente con le attività finanziarie, tipiche delle banche del Nord, non mi pare un'assunzione di responsabilità adeguata. Il voto capitario ha certo nascosto clientelismi e tendenze alla conservazione. Su questo la Banca d'Italia ha ragione. Taluni presidenti - lo ha ricordato la senatrice Ricchiuti - hanno avuto perfino problemi legali. Ma la stabilità in altre popolari ha prodotto gestioni assai positive. Ricordo il *tour* che feci in campagna elettorale in Valtellina a questo proposito. D'altra parte, vorrei ricordare - per esempio - che la Bipop, una delle popolari più grandi ai suoi tempi, si trasformò in SpA e diede luogo poi a tutte quelle contestazioni che vennero mosse alla Popolare di Milano, che era rimasta SpA. Cancellando il voto capitario - lo dobbiamo sapere - mettiamo in vendita le popolari maggiori e i compratori saranno esteri. L'asta per l'Istituto centrale delle banche popolari, in atto in questi giorni, è il prologo del fenomeno.

Preso atto dell'irremovibilità del Governo e degli orientamenti della Banca d'Italia, avevo suggerito non già una resistenza inconcludente a difesa del voto capitario, ma l'introduzione di limiti stringenti al diritto di voto, revocabili

Bastano quattro furbetti del quartierino che rastrellano e si mettono d'accordo per conto terzi e il gioco è fatto. È già accaduto alla BNL nel 2005. Di più, il 5 per cento a tempo è meno protettivo del 5 per cento senza scadenze di Unicredit. Perché questo doppio regime? Il vice ministro Baretta in Commissione ci ha detto che questo limite

che ha la forza e il consenso che dice di avere, potrà inserire negli statuti, nei prossimi mesi, il limite del 2-3

le banche popolari a diventare *public company* contendibili sul mercato, ha già prodotto e sta per produrre alcune conseguenze facilmente immaginabili. L'osservazione di quanto sta avvenendo realmente aiuta più di qualsiasi altro ragionamento, discorso o audizione a capire la portata della decisione presa dal Governo. La prima evidentissima conseguenza è che oggi la prima linea del *management*, inclusi gli amministratori delegati di una parte così rilevante del sistema bancario italiano, è impegnata in discussioni, negoziazioni e trattative per decidere chi si fonderà e come. In pratica, in una fase economica che definire delicata è poco, tra venti di guerra e ipotesi di spaccatura dell'euro, il *management*, invece di occuparsi di crediti, sarà in tutte altre faccende affaccendato e siamo certi che ciò non sia indifferente per imprese e correntisti. La seconda conseguenza è che sul mercato si è scatenata la speculazione peggiore, quella più antipatica e di breve periodo. Non si capisce davvero chi possa credere che l'*exploit* delle banche popolari possa essere legato ad ipotesi di creazione di valore di lungo periodo, su cui è lecito dubitare, che sono sicuramente, in ogni caso, indimostrabili. L'investitore di lungo periodo ha due questioni principali da risolvere prima di investire su una banca regionale italiana. La prima e più importante è quella sulle prospettive economiche italiane; la seconda è quella sulla solidità degli attivi. La trasformazione in società per azioni delle popolari non ha nessun impatto sulla prima questione; mentre per la seconda è davvero impossibile non contemplare nella propria analisi gli esempi fulgidissimi che ci hanno dato alcune *public company* "squotate"e tenute in grandissima considerazione da agenzie di *rating* come Lehman Brothers, Northern Rock, Bear Stearns, passando per quelle nazionalizzate in Europa. È più comprensibile, verificabile e controllabile un investimento in una banca che sostanzialmente, e persino con qualche svarione, investe sicuramente e principalmente nel territorio in cui ha le filiali, o in una che naviga le agitatissime acque dei mercati finanziari globali, magari con strumenti finanziari complessi e opachi? Nessun investitore, insomma,

Queste ultime, però, non sono fatte con i modi e i tempi degli italiani, che ancora magari si fanno scrupolo di lasciare a casa la gente da un giorno all'altro, e i tempi degli investitori globali, che devono rientrare il prima possibile dall'investimento. Questo è quanto c'è sul tavolo, al di là dei ragionamenti riportati da certi giornali sui benefici delle *public company*, guardati con un misto di tenerezza e divertimento da quelli che comprano per fare *performance* e hanno capito immediatamente che c'è solo e soltanto tantissimo valore finanziario da creare nel breve. La terza conseguenza è che un terzo del sistema bancario nostrano rimarrà quotato senza alcun azionista di controllo stabile italiano di lungo periodo. È evidente e palese che questa fetta del sistema finanziario verrà consegnata e messa sull'altare dei mercati finanziari globali e di investitori che gestiscono masse per centinaia di miliardi di euro, senza nessun tipo di mediazione. A questo riguardo ci sono due posizioni. La prima è quella di chi pensa che i mercati finanziari globali siano una forma neutra e positiva, che costringe a massimizzare il valore per gli azionisti e, quindi, è benefica in quanto tale. La seconda è quella di chi guarda con sospetto il mercato lasciato a se stesso, in cui logiche di massimizzazione del profitto di breve periodo sono irresistibili per il percettore di *bonus* e salari annuali, ma sono fuori dal grafico rispetto ad una persona normale, per la quale qualsiasi considerazione di medio periodo o di beneficio per l'economia, per non parlare del bene comune, è solo un ragionamento lunare più che incomprensibile. Chi vogliamo che controlli i risparmi e i prestiti alle imprese? Di più, la ripresa che si vuole è quella dei corsi azionari per i pochi fortunati che beneficiano delle grandi svendite o è la ripresa dell'economia per tutti? Questo provvedimento ha poi al suo interno anche un elemento straordinariamente irrazionale, che è il perimetro della riforma stessa, la famosa soglia degli 8 miliardi di euro prevista dal Governo, a mio avviso - irrazionale e persino incoerente con le sue finalità. Qualcuno ci dovrebbe dire atti perché questa riforma dovrebbe interessare solo le banche popolari con un attivo superiore agli miliardi di euro piuttosto che tutte. Qualcuno altresì ci dovrebbe dire perché il riferimento è all'attivo patrimoniale e non al patrimonio netto, magari al netto degli ammortamenti. Ritengo che la soglia degli 8 miliardi di euro non sia rappresentativa di alcun criterio né industriale né di vigilanza. Secondo me, l'identificazione di una soglia legata alla dimensione dell'attivo scoraggerà il consolidamento tra le banche popolari più piccole, che potrebbero essere indotte a non percorrere ipotesi di sviluppo e razionalizzazione, magari arrivando a ridurre le erogazioni creditizie, se questo dovesse determinare il superamento della soglia. Nessuno in realtà ci ha spiegato perché 8 miliardi di euro. O forse è talmente facile capirlo che non c'è bisogno di spiegazioni? Perché 8 miliardi di euro? Perché ci doveva rientrare qualcuno e non qualcun altro? Perché non tutti? Domande che finora non hanno avuto risposta dal Governo. Secondo degli studi di provenienza europea, si ritiene che il massimo dell'efficienza al crescere della dimensione di realizzi con un attivo intorno ai 20 miliardi di euro, mentre esiste un altro parametro di riferimento che avrebbe potuto essere quello relativo ai famosi 30 miliardi di euro, cioè la soglia che identifica gli istituti soggetti alla vigilanza diretta della BCE. E allora spiegateci perché 8 miliardi di euro. Devo ricordare, per aver fatto parte della Commissione economica del Parlamento europeo per molti anni, che la discussione sostenuta - per esempio - dal Governo tedesco, dai parlamentari tedeschi e dalla stessa cancelliera Merkel sulle *Landeskassen-Sparkassen* è sempre stata incentrata sulla soglia di vigilanza, i 30 miliardi, e in ogni caso quelle banche sono state difese con qualche successo. Torno dunque a chiedere: perché proprio 8 miliardi di euro? è poi la questione del diritto di recesso. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 di questo decreto-legge interviene sul diritto di recesso, per evitare che il rimborso delle azioni possa riflettersi negativamente sulla computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primarie della banca. Questo presenta vere criticità: si attribuisce alla Banca d'Italia una potestà generale in relazione a tutte le ipotesi di recesso. Non si capisce perché le stesse esigenze che sottendono alla soprarichiamata disposizione del decreto-legge non debbano applicarsi a tutti i soggetti sottoposti ad un regime di vigilanza potenziale. Questo decreto-legge consente, cioè, alla Banca d'Italia di sterilizzare non il diritto di recesso in sé, ma quello al rimborso delle azioni in caso di recesso, creando disparità a seconda che la banca sia quotata o meno E parliamo anche delle conseguenze per la mancata trasformazione. Tali trasformazioni possono variare secondo una gradazione che arriva fino alla messa in liquidazione dell'ente. Così facendo, si attribuisce al regolatore un potere che non ha alcuna mitigazione dal punto di vista della discrezionalità tecnica. La trasformazione obbligatoria avrebbe potuto essere configurata come *extrema ratio* nel caso in cui le banche popolari non avessero seguito un percorso di riforma della *governance*, secondo le direttive condivise caso per caso con la vigilanza. Questo decreto-legge, oltre alle ripercussioni sulle economie locali, andrà a distruggere il rapporto che dura ormai da oltre 150 anni tra banche popolari, famiglie e piccole e medie imprese, che rappresentano il vero motore economico dell'Italia. E qui veniamo al punto, su cui concludo, ad uno Stato e ad un Governo che fanno qualcosa per cambiare gli assetti e le *governance* di ciò che tiene in piedi quella che chiamiamo la sussidiarietà di un Paese (cioè il fatto che lo Stato riconosca sempre prima e comunque ciò che i cittadini fanno nell'iniziativa economica ed anche creditizia per venire incontro alle domande ed ai bisogni

Il riflesso peggiore di questo decreto-legge è che incrina questo rapporto tra le istituzioni e le comunità locali e, così facendo, crea le premesse per il dissolvimento di quella vita sociale e di quel "più società" che fanno bene allo Stato e sono stati la forza vera ed il motore di una qualsivoglia ripresa economica. Torno a chiedere: la ripresa che si vuole è quella dei pochi che avranno beneficio dalla gestione di azioni o quella dell'economia tutta, per la quale varrebbe la pena che le banche popolari possano autoriformarsi, senza essere riformate obbligatoriamente, per veder cancellata la propria storia? Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti della Scuola secondaria di primo grado «Istituto Mazzini-De Cesare» di Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Signor Presidente, oggi, 24 marzo, ricorre l'anniversario del massacro delle Fosse Ardeatine. Come ogni anno, la commemorazione si tiene al Mausoleo di Roma, alla presenza delle alte cariche dello Stato e numerosi componenti del Governo.

Con tale atto, diretto al ministro dell'interno Angelino Alfano, al quale abbiamo rivolto vari solleciti, chiedevo di riferire riguardo alla celebrazione dei funerali del carnefice delle Fosse Ardeatine, il generale nazista Erich Priebke, disposta all'epoca dal prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, nella cittadina di Albano Laziale, che purtroppo, come altre dei Castelli, ha avuto a piangere diverse vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Tale decisione del prefetto provocò all'epoca scontri, tensioni e feriti proprio

manifestanti ai quali va tutta la mia solidarietà, chi ha la responsabilità di questo pericoloso atto, che è stato una celebrazione fascista in piena regola, deve ancora venire a riferire in Aula sul caso. Invito quindi il Presidente, anche se un po' distratto dal suo telefonino, a sollecitare il ministro Alfano e i miei colleghi, che si professano democratici e antifascisti, a a sottoscrivere questo atto e sollecitare il Governo a prendere una posizione inequivocabile, e non solo di forma, sulla questione dei funerali di Erich Priebke. Presidente, colleghi, intervengo in merito ai fatti accaduti ieri pomeriggio nella città di Brescia. Mi riferisco al funzionario di polizia incaricato di mantenere l'ordine pubblico,

Ho potuto quindi verificare con i miei occhi le criticità che affliggono la struttura. La più evidente e paradossale è proprio la mancanza di lavoro: si tratta di una casa lavoro soltanto di nome, perché di fatto il lavoro non esiste e quindi non esiste il percorso di riabilitazione per reintegrare gli internati nella società. Per il personale del carcere di Vasto - perché di carcere si tratta - di lavoro invece ce n'è pure troppo. Attualmente sono in servizio 105 unità della Polizia penitenziaria, mentre la stessa amministrazione ha fissato a 125 unità l'organico minimo necessario. Teniamo inoltre presente che, fra detenuti e internati, la cosiddetta Casa lavoro di Vasto è cronicamente affollata oltre il limite della sua capienza. Nonostante questo, invece di assumere nuovi dipendenti e far finalmente partire opportunità di lavoro per gli internati dopo due anni di ozio,

Si tratta quindi di pretendere da 105 persone di lavorare come se fossero 140. Fra l'altro, non parliamo di giovanotti: non c'è ricambio da molto tempo e l'età media degli agenti è piuttosto alta. Possiamo solo immaginare quanto sia logorante, nel corso degli anni, un lavoro di responsabilità a contatto quotidiano con persone fortemente disagiate, spesso con problemi di salute sia fisica che psicologica. Di fronte al precipitare di una situazione già compromessa in partenza, le organizzazioni sindacali di categoria hanno scritto una lettera indirizzata a vari destinatari, tra cui anche il sottoscritto, dichiarando lo stato di agitazione e la possibilità di forme di protesta più eclatanti. Mi sono quindi sentito in dovere di far presente il problema a quest'Assemblea e di sottolineare che non si tratta di un caso isolato, ma nella norma nel nostro Paese. Le nostre Forze dell'ordine sono state abbandonate ed umiliate da Renzi e dai suoi predecessori. Quando il Presidente del Consiglio sostiene che cinque Forze di polizia sono troppe e parla di fusioni per risparmiare ed evitare sprechi, dimentica di dire che nessuno in Europa spende meno di noi in politiche di sicurezza. In proporzione al PIL, la Spagna investe 10 volte tanto; Francia e Germania addirittura 15. Quindi permettetemi di concludere con una domanda populista: perché in Italia non ci sono soldi per assumere qualche agente penitenziario in più, mentre ci sono soldi in abbondanza per pagare vitalizi ai politici condannati per mafia e corruzione?